"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

che sale agli onori della cronaca. Il punto è un altro: il Parlamento vuole affrontare in maniera efficace e con strumenti efficaci il problema della corruzione nel nostro Paese oppure no? Di questo dobbiamo discutere e su questo dobbiamo votare tra poco.

Oggi quella legge porta il nome del presidente del Senato ed è un alibi per i partiti di maggioranza per dire di aver fatto qualcosa. Io - è una mia opinione - toglierei il mio nome, proprio per non essere strumentalizzato da questo punto di vista. In televisione questa è la posizione: abbiamo portato avanti delle riforme. No, 1.400 giorni sono stati necessari per smantellare quelle riforme. Basta fare un confronto tra la legge approvata e il disegno di legge del Partito Democratico - non parlo di quello del Movimento 5 Stelle - e vi accorgerete che in questo Parlamento non c'è alcuna volontà

È un problema che si porta via decine di miliardi ogni anno. I rapporti annuali della Guardia di finanza sono impietosi. Basti pensare che un terzo degli appalti pubblici controllati sono stati assegnati illecitamente, per non parlare poi del rinnovo delle concessioni autostradali senza gara pubblica, come nel caso della A4 Padova-Brescia, che non è stata messa a gara per consentire al concessionario privato di privato di vendere la concessionaria e realizzare plusvalenze per miliardi che sono denari pubblici trasferiti a privati. Magari tra qualche anno conosceremo le ragioni vere di questa operazione. Il problema non è solo economico. La corruzione si porta via posti di lavoro e senza la corruzione la mafia non sarebbe così forte. forte. Non è tanto la mafia che alimenta la corruzione; è la corruzione che crea un ambiente ideale per lo sviluppo della criminalità organizzata nel nostro Paese. Venendo al contenuto del disegno di legge, di cui chiediamo la trattazione di urgenza, credo dovremmo fare particolare attenzione a questi punti. "un condannato per corruzione dovrebbe essere escluso dal giro dei lavori pubblici per sempre". In secondo luogo, "tu che hai corrotto o concusso qualcuno, mi fai la cortesia di non mettere più piede negli appalti pubblici". "ci vuole il DASPO per i politici che tradiscono la fiducia dei cittadini". "Il punto centrale è garantire che chi viene condannato non torni più a occuparsi della cosa pubblica". E ancora, ma potrei continuare - "fanno il DASPO ai tifosi, va fatto il DASPO ai politici che prendono tangenti: mai più!" Immagino che qualcuno abbia sicuramente capito che non sono frasi mie, ma di Matteo Renzi, pronunciate durante il suo intervento a Milano, a Forlì e persino a margine del G7 di Lussemburgo. Il DASPO, per chi non lo sapesse, è una misura prevista dalla legge che consente al questore di vietare, al tifoso ritenuto pericoloso, l'accesso alle manifestazioni sportive. Secondo Renzi bisognerebbe garantire che un condannato per corruzione venga allontanato per sempre dalla cosa pubblica, un'interdizione perpetua, insomma. il dichiarato il *Premier*. Addirittura, sempre secondo Renzi, i politici già indagati per aver preso tangenti andrebbero ulteriormente indagati per alto tradimento allo Stato per aver violato il mandato su cui hanno giurato.

In Commissione giustizia Partito Democratico e maggioranza hanno già respinto un emendamento che prevedeva l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Questo naturalmente in caso di Si trattava di un emendamento che avrebbe interdetto ed allontanato sul serio dalla cosa pubblica tutti i condannati per i reati di concussione, corruzione e peculato. L'emendamento proponeva le parole e le intenzioni del Presidente del Consiglio. Allontanare definitivamente i ladri dalla pubblica amministrazione per non concedere più occasione di reiterare lo stesso reato, cosa che avviene quotidianamente. Bene, è lo stesso emendamento che abbiamo presentato sotto forma di disegno di legge. Cantone ha formulato una proposta analoga, così sintetizzata: prendi una tangente, perdi l'appalto. E noi aggiungiamo: e con la pubblica amministrazione non ci lavori più. Anche il Consiglio superiore della magistratura ha assunto la medesima posizione. A proposito di corruzione, ha infatti dichiarato: «Sul piano sanzionatorio andrebbe ripensato l'intero sistema delle pene accessorie, prevedendo come obbligatoria l'interdizione perpetua per ogni fattispecie corruttiva». In conclusione, noi siamo qui a chiedere di trattare con urgenza un provvedimento più volte invocato dal *Premier*, a reti unificate e in eurovisione, auspicato dai magistrati, da chi combatte la corruzione e da 60 milioni di cittadini onesti. Ma se la proposta non dovesse trovare accoglimento, mi permetto di suggerire un'altra soluzione, altrettanto democratica, per far guarire l'Italia dalla corruzione: torniamo subito alle urne e diamo ai cittadini la possibilità di ripulire questo Parlamento, che evidentemente non sta dando prova di pulire se stesso! *(Applausi

Presidente, a questa richiesta non vogliamo dare una risposta liquidatoria,

La corruzione è il problema dei problemi del nostro Paese. Negare o minimizzare fa male ai nostri cittadini, allo sviluppo e alla democrazia della nostra società. società. È una sfida aperta. Con onestà intellettuale, però, nessuno può negare che in questa legislatura si sia fatto un lavoro mai fatto prima. Mai, nel Parlamento italiano, si erano approvate leggi, misure e strumenti nella lotta alle mafie e alla corruzione, che oggi corrispondono, come non mai, a due facce diverse di una stessa medaglia. Perché questo, signora Presidente? Ricordo ai colleghi che mai, nel nostro Paese, si era costruita un'agenzia come l'ANAC, con veri poteri. Adesso essa si sta adeguando per dotarsi di una struttura potente e in grado di svolgere tutte le funzioni che il Parlamento e il Governo le hanno assegnato. Presidente, per anni abbiamo lottato per avere una legge sul falso in bilancio. Adesso c'è. E così è sull'autoriciclaggio. Ricordo ai colleghi che proprio qui al Senato, nella legge di riforma degli appalti, abbiamo inserito nella delega al Governo delle misure che vanno proprio nella direzione di allontanare per sempre le imprese che pagano il pizzo e che partecipano alla corruzione. E così per i funzionari pubblici che nel sistema degli appalti giocano utilizzando la corruzione.

proprio da qui al Senato è partito un aumento delle pene nella lotta alla corruzione senza precedenti. Oggi, grazie a quell'aumento di pena, chi utilizza la corruzione non può più ricorrere all'*escamotage* della prescrizione. Ma non basta, cari colleghi. Abbiamo anche inserito una norma che impedisce il ricorso al patteggiamento per chi corrompe.

ecco perché mi rivolgo direttamente ai colleghi. Vi ricordo che abbiamo due misure in corso di approvazione, due misure che un ramo del Parlamento ha già varato. Mi riferisco alla riforma del processo penale, dove sono inserite delle norme che vanno a colpire la corruzione. Abbiamo introdotto un aumento della pena - cosa impensabile, che ci ha diviso e che ha anche lacerato il lavoro del Parlamento - per quanto riguarda l'articolo 416-*ter*, che è il reato più odioso, perché si riferisce allo scambio politico-elettorale.

la possibilità di utilizzare uno strumento, che il collega Cappelletti non ha indicato, che forse è il più potente di tutti e che gli esperti alla lotta alla mafia conoscono bene: la misura di prevenzione patrimoniale e personale da applicare a reati di corruzione.

Si vuol fare di più, si vuol ricorrere, come noi del Partito Democratico proponevamo, al DASPO, all'agente sotto copertura (questa norma era inserita nel testo Grasso). Siamo pronti, colleghi, ma la via più veloce non è quella di iniziare un nuovo *iter* legislativo. Ecco perché lì si manifesta l'ipocrisia e anche uno strumento contraddittorio con l'idea che si ha di accelerare i tempi e di affrontare questo nodo, perché la Camera ha già approvato che vanno in questa direzione in ben due testi e la Commissione giustizia è già al lavoro: lì è il luogo in cui misurarsi con queste sfide.

il suo persecutore, l'inflessibile ispettore che alla fine si suicida. Mi sono messo nei panni di uno spettatore di un film di questo genere

bisognerebbe mettere in galera i corrotti, ma anche quelli che dovrebbero mettere in galera i corrotti, cioè la Polizia, i Carabinieri e la Guardia di finanza: tutti in carcere. Per fortuna le cose non stanno così. La corruzione non si combatte con i proclami; intanto la si contrasta con un'opera di educazione alla legalità - che è importantissima - già nelle piccole cose, a cominciare dai favori, dai compiti che vengono copiati a scuola, come scriveva il «Corriere della sera», da una mentalità che considera furbo chi prende scorciatoie. Poi si combatte facendo fare ai magistrati, quelli veri e seri, il loro mestiere. Ad esempio, in Veneto un magistrato che si chiama Nordio, che la pensa esattamente come me sui metodi per combattere la corruzione, in pochi mesi ha smantellato una rete corruttiva senza aspettare i ventun anni della prescrizione; ha già condannato tutti i responsabili compresi i politici che erano a capo di quella rete (facendo indagini serie,

è tutto il mio dissenso con il collega Lumia): «Sì, la lotta alla mafia la facciamo anche alle imprese, andiamo ai sequestri preventivi sulla base dei sospetti?». Altro che commissario Javert, stiamo andando su una strada

che per avere quello che un cittadino o un'impresa doveva avere in maniera trasparente o diretta occorrevano invece 56 passaggi amministrativi e si complicavano sempre più i meccanismi, per cui chi si confrontava con queste difficoltà cercava le scorciatoie? se il rapporto con la pubblica amministrazione fosse chiaro, limpido, con tempi certi, se si sapesse chi ha diritto a cosa in tempi sicuri e non complicassimo il tutto, come stiamo facendo ovunque con la moltiplicazione delle procedure burocratiche e dei controlli. Chi dice che il controllore non sia corrotto come il controllato? Chi dice che i 20 passaggi

e in effetti lo ha fatto. Un conto è quando ci riferiamo a casi concreti, un altro quando si fanno generalizzazioni che comportano questa coazione a ripetere.

visto che gli apprendisti stregoni finiscono sempre impiccati all'albero e alla corda cui pensano di impiccare gli altri, considerate che più l'inchiesta è sbagliata fin dall'inizio, più l'arresto è ingiustificato, meno elementi

perché non venga dimostrato che l'ipotesi accusatoria iniziale era infondata. Non entro nel merito delle proposte che vedremo in Commissione, ma invito tutto il Parlamento a non seguire i giacobini, che hanno distrutto la Francia rivoluzionaria

alla corruzione con molto pragmatismo, come ho detto prima, innanzitutto ricorrendo ad un grande strumento nazionale, educativo, culturale, nella scuola e ovunque

come riconoscono i tribunali (quando si arriva in tribunale), il Consiglio di Stato (quando si arriva in Consiglio di Stato) o il Ministero dell'interno (quando si arriva al Ministero dell'interno); ma è troppo tardi, perché il danno in quel momento è già stato fatto.

questi temi per interessi propri. Il mio è solo un invito al Parlamento alla prudenza e alla saggezza quando si legifera in queste materie. (MpA))*. Signora Presidente, farò un intervento molto breve per dire che il voto del Gruppo AL-A è contrario.

ci sono i difensori della giustizia, mentre tutti coloro i quali non la difendono sono paradigmaticamente dei potenziali mascalzoni. Io invece ho imparato, nella mia - ahimè - lunga vita, a conoscere molti mascalzoni che non erano moralisti;

perché, sia in sede civile, sia in sede penale, abbiamo processi che durano in eterno. Io immagino un imprenditore, che dovendo già affrontare i rischi dell'impresa,

della giustizia penale perché ci ripeteremmo, ma voglio solamente soffermare l'attenzione sulla parte civile, su quanto dura un contenzioso tra due persone. Abbiamo provato, con l'istituzione del patteggiamento, della transazione tra le parti, ad alleggerire questo carico, ma purtroppo non ci siamo riusciti.

dobbiamo affrontare organicamente il problema senza avere la presunzione di essere moralmente migliori degli altri. Nello Stato di diritto la morale risiede nella legge e siamo tutti quanti sottoposti alla legge e in questo contesto, coloro che ci hanno preceduto in queste Aule vollero modificare la procedura stabilendo che la prova si forma nel dibattimento. Siamo passati dal rito inquisitorio, dove il cittadino aspettava le grazie del giudice istruttore per sapere se era o no inquisito, ad un istituto di maggiore garanzia per i cittadini, non per i politici. L'avviso di garanzia informa l'imputato che è stato avviato un procedimento a suo carico e se la prova si forma nel dibattimento, nell'antitesi tra accusa e difesa, gli avvisi di garanzia sono tali; non sono sentenze di colpevolezza, non sono la clava attraverso la quale una forza politica può tentare di delegittimare, criminalizzare e infangare un'altra forza politica. Altrimenti vivremmo in uno Stato di polizia,

perché se amiamo la giustizia dobbiamo stare attenti agli zelatori della giustizia, a coloro che la usano per sostenere il vuoto pneumatico che hanno in testa, esibendo la giustizia e l'esasperazione del concetto giustizialista come motivo ontologico della loro presenza.

società. Mi permetto di ripetere in quest'Aula quello che Robespierre disse alla marchesa di Condorcet, la quale contestava finanche Robespierre, nonostante la politica del terrore. Allorquando, alzandosi nell'Assemblea costituente, ella disse, vicino a Robespierre: «Se lei fosse mio marito, le propinerei del tè avvelenato»,

Signora Presidente, ho chiesto di intervenire perché dopo gli interventi degli esponenti del Partito Democratico, di A-LA e del senatore Giovanardi, ritenevo opportuno, e utile per tutta l'Assemblea, chiarire un paio di punti. Intanto prendiamo atto che secondo la maggioranza, da quanto si evince dall'intervento del senatore Lumia, di fatto la proposta del disegno di legge a prima firma Cappelletti che vuole estendere il cosiddetto DASPO ad altre ipotesi di reato viene accettata perché, sempre secondo il senatore Lumia, la maggioranza, il Parlamento e il Governo hanno già operato sufficientemente in materia di corruzione lo scorso anno con la legge n. 69, pertanto non c'è bisogno di ulteriori misure volte a scoraggiare il fenomeno corruttivo. Peraltro, il senatore Lumia ha dimenticato che il collega Cappelletti aveva citato letteralmente l'intervento del Presidente del Consiglio quando quando inneggiava al DASPO per i corrotti: questa contraddizione si staglia chiarissima all'orizzonte. Inoltre, che sia la Commissione giustizia il luogo

interdittive che già sono previste oggi. Se prendete il disegno di legge n. 1954, all'articolo 1 vedrete una proposta di modifica dell'articolo 317-*bis* del codice penale, che già oggi prevede che, in caso di condanna definitiva per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, ne consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua a contrattare con la pubblica amministrazione. Il nostro disegno di legge vuole semplicemente estendere questa misura anche ai casi di sentenza di condanna per corruzione per l'esercizio della funzione. Si tratta dell'articolo 318 del codice penale, la cui pena massima è stata aumentata l'anno scorso fino a sei anni di reclusione - lo ricordo - proprio grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle,

per un atto del proprio ufficio. A noi sembra - e riteniamo sembri anche agli italiani - incomprensibile questo ostinarsi a non voler estendere anche a queste fattispecie di reato la

che si vuole rincorrere il moralismo, con argomentazioni sostenute anche dal senatore D'Anna, che francamente ha dedotto argomentazioni che non c'entrano nulla con il disegno di legge di cui stiamo parlando. Qui non si parla di prescrizione, non si

ascoltata - da parte della forze politiche presenti in quest'Assemblea: siamo d'accordo o no ad estendere il cosiddetto DASPO, oltre alle ipotesi già previste oggi dall'articolo 317-*bis* del codice penale, anche ai casi di corruzione, *ex* articolo 318, e di induzione indebita a dare o promettere utilità, *ex* articolo 319-*quater* anche estendendola all'incaricato di un pubblico servizio? Questo è quello che il disegno di legge propone; è inutile allargare le argomentazioni a questioni filosofiche o moraleggianti. Mettiamo da parte ogni intento polemico o e chiediamo all'Aula, ai partiti della maggioranza e dell'opposizione: siete d'accordo sì o no - e facciamolo sapere agli italiani - ad estendere l'incapacità a contrarre, l'incandidabilità per le pubbliche funzioni e l'incapacità a ricoprire incarichi pubblici, una volta per tutte, anche a questi casi di corruzione? Sì o no? Poi gli italiani valuteranno se sono proposte alla Robespierre, se sono proposte ragionevoli e necessarie oppure no.

Cari colleghi che protestate, il Regolamento dà al Presidente

del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*** La relatrice, senatrice Puglisi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi Signora Presidente, onorevoli colleghi, il testo che discutiamo oggi in Assemblea è un decreto-legge che interviene

Per prima cosa esso contiene disposizioni per assicurare la prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro degli edifici scolastici e lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. Si tratta di 64 milioni di euro per il 2016 per garantire la prosecuzione del piano scuole belle, che consiste in un piano di interventi per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, avviato dal Governo nel 2014, nell'ambito del più vasto piano per l'edilizia scolastica, che include un piano triennale di 3.700 milioni di euro nel triennio, per scuole sicure e scuole nuove. Quella dell'utilizzo degli ex lavoratori socialmente utili (LSU) nell'ambito del piano scuole belle è una vicenda che nasce da lontano. Nel 1999, infatti, lo Stato subentra agli enti locali nei rapporti di lavoro dipendente con il personale scolastico non docente, tra i quali figuravano all'epoca i collaboratori scolastici (per la maggioranza provenienti dal bacino degli ex lavoratori socialmente utili) e, tra il 2000 e il 2001, lo Stato subentra anche nei contratti di servizio con le imprese coinvolte, per una spesa annua di circa 624 milioni Nel 2009, il Governo Berlusconi avvia un piano di riduzione della spesa per la pulizia delle scuole, che porta una riduzione di circa il 10 Nel 2011 l'importo complessivo degli acquisti viene ulteriormente ridotto mediante un accordo con le imprese a 390 milioni di Oggi, circa 5.000 scuole coprono le proprie esigenze di pulizia e altri servizi ausiliari, come la vigilanza degli alunni o la sorveglianza degli accessi, esclusivamente mediante ricorso a collaboratori scolastici dipendenti statali. Altre 3.600 scuole circa, invece, acquistano i relativi servizi da imprese. Nel 2013 è stato introdotto un limite di spesa per l'acquisto dei servizi in questione, ponendolo pari a quanto si spenderebbe per svolgerli mediante esclusivo ricorso al personale dipendente, ovvero, vista la scopertura di circa 11.800 posti di collaboratore scolastico, pari a 300 milioni di euro l'anno. Contemporaneamente, la Consip ha bandito un'apposita gara, che è stata aggiudicata ed attivata il 1° gennaio 2014. Questa gara, divisa in 13 lotti (corrispondenti per lo più al livello regionale; in alcuni casi interregionale) è stata aggiudicata dappertutto, con scadenza il 31 dicembre 31 dicembre del 2016, tranne in Sicilia e Campania, in cui sono intervenuti contenziosi (tuttora in essere davanti al giudice amministrativo e, nel caso della Campania, davanti alla Corte di giustizia europea) tra l'aggiudicatario provvisorio e i controinteressati. Quindi, in queste due Regioni la gara è stata effettuata dalla Consip, ma ancora non è stata aggiudicata. Soltanto recentemente, come comunicato dalla Consip, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato del 17 marzo del 2016, si è giunti ad una soluzione del contenzioso per il lotto relativo alla Sicilia ed è in corso la stipula del contratto tra la Consip e l'impresa aggiudicataria, con la conseguente imminente attivazione della convenzione. Naturalmente la riduzione degli importi destinati ai servizi di pulizia e i risparmi derivanti dal ricorso alla gara Consip non poteva non avere effetti sulla continuità occupazionale e reddituale dei dipendenti delle imprese, ex LSU, che pur ridottisi di numero nel tempo - dai poco più di 24.000 del 2000 ai 18.148 del 2016, dislocati soprattutto al Sud - rimanevano troppi per trovare tutti integralmente impiego nell'ambito dei contratti con le scuole per i servizi

aggiudicatari degli appalti Consip, il Governo ha trovato una soluzione per i 18.000 lavoratori, ex LSU, formandoli per prestare servizio per lavori di manutenzione degli ambienti scolastici, migliorando la vivibilità delle classi e degli ambienti comuni. Gli interventi sono stati inseriti nel piano straordinario scuole belle per il mantenimento ed il ripristino delle funzionalità e il decoro degli edifici scolastici pubblici, che rientra nel più ampio programma di Governo dedicato al miglioramento delle condizioni e all'efficientamento dell'edilizia scolastica Con il piano scuole belle, che ha comportato un investimento di 450 milioni di euro dal 1° luglio 2014 al 1° aprile 2016, non solo si è data una risposta all'occupazione, ma si è riusciti a realizzare 15.996 interventi di decoro e di manutenzione delle scuole. Con questo decreto viene poi finanziata con 3 milioni di euro la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) che, dopo il parere favorevole dell'ANVUR, diventa stabilmente istituto universitario La Scuola, inizialmente attivata in via sperimentale dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel dopo-terremoto, nasce per rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo con la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, per realizzare un polo di eccellenza internazionale, grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, e favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base. Quindi, grazie a questa stabilizzazione, si può procedere al reclutamento di personale. Ma questo provvedimento interviene su molti altri punti davvero utili soprattutto alla scuola, dopo anni di tagli, per continuare a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli insegnanti e di studio degli Prima di tutto contiene lo stanziamento necessario a raddoppiare i compensi dei commissari del concorso scuola (che è in corso in queste in queste settimane), così come promesso dal Presidente del Consiglio. Assicura inoltre il pagamento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze brevi o saltuarie degli insegnanti entro trenta giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento. riferimento. Il mancato rispetto dei termini, che non è novità di questo anno ma che purtroppo era cronico, diventa fonte di responsabilità dirigenziale qualora le cause del ritardo siano imputabili al personale MIUR o MEF. Al personale docente e ATA sarà anche assegnato un codice identificativo per facilitare l'assegnazione delle partite stipendiali. i 100.000 docenti assunti con il piano straordinario della buona scuola e in generale tutti quelli di ruolo potranno chiedere per il prossimo anno scolastico, in deroga al vincolo triennale, assegnazione provvisoria interprovinciale sui posti residuali di diritto eventualmente rimasti dopo mobilità e e assunzioni in ruolo, ma anche, per la prima volta, su organico di fatto, allargando quindi di molto l'opportunità di restare o tornare a lavorare vicino ai propri cari. Con questa misura non si generano - sia chiaro! - maggiori o minori supplenze, semplicemente cambia il luogo dove si nomina il supplente. Questo permetterà di attenuare gli effetti dello spostamento dei docenti verso Nord, che in quest'anno scolastico, pur entrati in ruolo lontano da casa, sono potuti rimanere, grazie alla norma della legge n. 107 del 2015, che consentiva la permanenza sulla supplenza se ottenuta prima dell'immissione in ruolo. Ancora una volta voglio ricordare a questa Assemblea che la mobilità degli insegnanti da Sud a Nord c'è sempre stata, a causa dei diversi *trend* demografici del Paese che vedono una popolazione scolastica in costante crescita in alcune Regioni del Centro Nord e in calo nel Mezzogiorno. Un'altra norma molto attesa, contenuta in questo decreto-legge, prevede il totale assorbimento, attraverso la mobilità interregionale volontaria, delle graduatorie di merito per la scuola dell'infanzia del concorso 2012; ancora, il rifinanziamento del fondo nel 2017 per il sostegno degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie con un contributo statale di 1.000 euro per alunno con disabilità frequentante, per un totale di 12,2 milioni. Questa - ci tengo a sottolinearlo - è una norma antidiscriminatoria nei confronti degli studenti con disabilità, per poter garantire anche alle loro famiglie il diritto alla libertà di scelta educativa. Delle due l'una: non possiamo accusare le scuole paritarie di non accogliere gli studenti con disabilità e poi non garantire, come hanno fatto altri Governi, le risorse per poterli accogliere. Sempre alle persone con disabilità è dedicata un'altra norma sull'ISEE che ne garantisce l'esclusione dal calcolo di ogni trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario erogato da enti pubblici. Inoltre, vi è un chiarimento molto importante - e atteso dagli studenti universitari - in quanto finalmente si esplicita che le aziende per il diritto allo studio debbono sottrarre dallo stesso ISEE le borse di studio percepite l'anno precedente dagli studenti capaci e meritevoli. Viene poi risolto il blocco dei corsi di specializzazione delle professioni non mediche che ha impedito a migliaia di giovani laureati magistrali (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) di potersi specializzare, con la sospensione della norma norma della legge n. 401 del 2000 nell'attuale formulazione, in attesa che il Ministero della salute ne stabilisca il fabbisogno per poter erogare le borse di studio. Infine, il Governo estende la *card* di 500 euro per i consumi culturali dei diciottenni alle ragazze e ai ragazzi Quindi, con un investimento di 290 milioni di euro saranno tutti i 576.953 diciottenni che risiedono nel nostro Paese, di cui 24.305 ragazzi e ragazze extra UE, a beneficiarne per assistere a rappresentazioni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Una misura di equità, civiltà e di vera inclusione, di piena cittadinanza per tutti i diciottenni, che fu annunciata da Matteo Renzi all'indomani della strage di Parigi in cui 93 ragazze e ragazzi - tra cui la nostra ricercatrice, Valeria Solesin -

bellezza e l'educazione che potremo davvero costruire davvero un'Europa di pace.

Senatore Buemi, stia calmo.

Presidente, solo per favorire il clima positivo che credo giovi a tutti, vorrei segnalare al collega Martelli

già così ben illustrato dalla relatrice, senatrice Puglisi. In particolare, viene assicurato il ripristino del decoro e della funzionalità di molte scuole grazie all'impegno del Governo,

scuole nuove, scuole sicure, insomma scuole belle. Il Ministero dell'istruzione ha stanziato altri 64 milioni di euro per tale proroga, che consente interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. Ma la scuola non dovrebbe essere all'attenzione generale e globale, colleghi? La scadenza del 1° aprile viene dunque prorogata di altri sette mesi grazie alle misure previste nel decreto-legge. Ciò consente di mantenere in servizio circa 18.000 addetti alle pulizie, di cui poco più di 12.000 ex LSU (lavoratori socialmente utili) utilizzati per piccoli interventi nella scuola, per la pulizia delle classi, la sorveglianza dei locali, per la vigilanza degli alunni e la piccola manutenzione. È difficilmente comprensibile che un'azione tempestiva e urgente a sostegno dell'occupazione di lavoratori in difficoltà abbia trovato tanta ostilità, un'ostilità strumentale, come è di tutta evidenza. Con lo stesso decreto-legge si autorizzano le scuole di Campania e Sicilia, dove la gara Consip non è partita, e le scuole del Lazio, dove scade, a continuare ad affidare, fino al 31 dicembre, i servizi di pulizia e ausiliari alle ditte che li hanno finora erogati. del 31 dicembre, peraltro, scadono anche le proroghe annuali delle convenzioni nelle altre regioni dove è decollato il sistema Consip. Sulla questione della pulizia ricordo che nel 2012 l'ex ministro Francesco Profumo decise di dare ordine al sistema e di acquistare i servizi a seguito di una gara Il MIUR è titolare di contratti di servizio per 620 milioni di euro, con ditte che impiegano l'equivalente di oltre 24.000 unità a tempo pieno, a fronte di una vacanza organica del doppio dei posti ATA, di 12.000 unità. Il programma scuole belle del Governo, per un importo complessivo di 450 milioni di euro l'anno, ha previsto e realizzato un totale di 17.815 interventi

tutto ciò di cui la scuola ha grande bisogno. In base alle risorse disponibili, le attività sarebbero durate fino a oggi e le aziende avrebbero dovuto poi licenziare gli operatori impegnati nelle attività di ripristino. Con il nuovo finanziamento il programma, invece, continuerà e si arriverà fino al mese di novembre. Nel periodo estivo il Governo si è detto disponibile ad accogliere eventuali richieste di cassa integrazione in deroga.

ripristinerà nelle scuole italiane la funzionalità; favorirà lo star bene a scuola degli studenti, dei docenti e degli operatori scolastici. però, competenza dei dirigenti pianificare gli interventi, in coordinamento con il consiglio di istituto e gli enti locali, e vigilare sull'attuazione del programma, sulla conduzione efficiente dei lavori, sulla qualità delle attività di manutenzione, sulla pulizia approfondita degli edifici.

di abbellimento e risanamento degli edifici, che gli studenti devono trovare curati, puliti e confortevoli tutto il giorno. Le scuole sono aperte tutto il giorno e, quindi, a maggior ragione c'è bisogno di servizi qualificati. Va dunque valorizzata e non sprecata questa grande occasione

la soluzione graduale a problemi come quello della mobilità e il rifinanziamento dei fondi per la disabilità. Insomma, il quadro complessivo si sta ricomponendo. I problemi strutturali e cronici del mondo della scuola sono in via di risoluzione ed è davvero una grande soddisfazione vivere dall'interno questo processo, vivere i suoi percorsi positivi per concretizzarlo e dare un contributo per ottimizzarlo. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere tutto il mio apprezzamento per l'istituzione della scuola di dottorato Gran Sasso Science Institute.

Sarà certamente una istituzione meritevole. A promuoverla sono i bravissimi scienziati dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, uno dei più prestigiosi tra gli enti di ricerca italiani. L'iniziativa si insedia nella generosa terra d'Abruzzo, vicino alla bella città dell'Aquila, contribuendo alla sua rinascita mediante la leva più efficace, che è l'investimento in conoscenza. Non posso però tacere le anomalie di metodo del provvedimento È curiosa l'istituzione per decreto-legge di una nuova università: è un'urgenza che deriva da una inadempienza ministeriale. Al Ministero sapevano bene che stavano per scadere i finanziamenti della sperimentazione e c'erano gli strumenti di programmazione adatti per prendere una decisione per tempo con procedure ordinarie. luogo, si finanzia una nuova università togliendo i soldi alle altre università e agli enti di ricerca: un altro taglio, oggi piccolo, ma che domani potrebbe crescere. È incredibile che la Commissione bilancio e il Ministero non abbiano fatto proiezioni nel tempo, prevedendo gli oneri di finanza pubblica del provvedimento Per evitare l'ennesimo taglio ho presentato l'emendamento 3.4, con il quale si intende finanziare la nuova università aquilana prendendo i soldi dal fondo dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), che abbonda di risorse fino al punto che non riesce a spendere i finanziamenti che riceve

81 della Costituzione, il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe attenersi solo a considerazioni sulla capienza dei capitoli, senza entrare nel merito delle politiche o - peggio ancora - privilegiare le sue preferenze o le sue amicizie. è notoriamente il cocco di casa a Via Venti Settembre: per tanti anni il direttore del Ministero è stato anche Presidente dell'istituto, in pieno conflitto di interessi. La stessa discrezionalità ha portato all'affidamento del progetto Human Technopole, finanziato con 80 milioni iniziali - ma si prevede di arrivare a 1,5 miliardi - che viene giustificato come una decisione *top-down*. Non c'è, però, alcuna ragione scientifica per non sottoporla a un confronto trasparente secondo le migliori esperienze internazionali. Ho sottoscritto l'ordine del giorno G2.1 della senatrice Cattaneo che spiega come fare, e lascio a lei l'onore di illustrarlo. Non c'è quindi alcuna giustificazione nell'assegnazione in esclusiva per legge a un solo soggetto del finanziamento, tanto meno nel caso dell'IIT che, svolgendo insieme attività di ricerca in proprio, non ha l'indipendenza necessaria per erogare finanziamenti ad altri: non può essere contemporaneamente un laboratorio e un'agenzia; non può essere giocatore e arbitro. Proprio con questo argomento alla fine degli anni Novanta si tolse al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) il potere di assegnare finanziamenti ad altri soggetti, perché già faceva ricerca nei suoi istituti. Allora si riteneva sbagliata la commistione di ruoli che oggi, invece, si ripropone in un soggetto privato che viene delegato completamente al salotto della finanza. Fu Tremonti a cancellare lo stanziamento per i fondi dei progetti di ricerca e a potenziare l'IIT. Aggiunse anche una regalia economica e simbolica di ciò che resta del patrimonio IRI dopo le privatizzazioni. Viene spontaneo un confronto fra le due fasi storiche: l'IIT ha preso dell'IRI tutti i vizi e nessuna virtù, ha rilanciato i vecchi vizi dei boiardi di Stato, che si dichiaravano soggetti pubblici quando ricevevano commesse senza gare, ma si comportavano da privati quando erogavano finanziamenti in cambio del consenso. Non ha rinnovato, però, la virtù che fu dell'IRI nella promozione dell'impresa di alta tecnologia, nonostante proprio questo fosse l'obiettivo definito nella legge istitutiva n. 326 Si è già speso oltre un miliardo di euro per la ricerca nella robotica umanoide, ma non è nata alcuna filiera produttiva capace di utilizzare quei risultati scientifici. Eppure - come dicevo - la gestione della Fondazione è stata delegata a esponenti del salotto della finanza e dell'impresa, che evidentemente si pavoneggiano con i soldi pubblici senza rischiare in proprio. Dopo un lungo ciclo siamo, quindi, tornati al punto di partenza, ma con minore libertà per la scienza. Come si è detto, la sovrapposizione dei ruoli tra Agenzia e laboratorio fu eliminata in un ente pubblico come il CNR e oggi viene, però, ricostituita in una Fondazione gestita dal dal salotto finanziario, senza trasparenza nelle procedure di assegnazione e senza garanzie per la comunità scientifica. È paradossale che, nelle sue prime dichiarazioni, il neo Presidente del CNR accetti questo sistema e si limiti a chiedere la sua parte: «Ci sarà una cabina di regia e noi parteciperemo», dichiara al «Corriere della Sera» l'8 marzo 2016, con una sudditanza che non sarebbe neppure immaginabile nel Max Planck tedesco o nel CNRS francese. C'è da augurarsi che il CNR ritrovi in futuro l'orgoglio della principale istituzione della ricerca italiana. La ricerca libera, quindi, è molto indebolita nel nostro Paese. Le risorse sono assegnate dal principe ai conti e ai vassalli, che le distribuiscono ai sudditi. È quasi scomparso il fondo FIRB, che finanziava negli enti i progetti dei ricercatori. Per ottenere risorse essi, oggi, devono sperare solo nelle trattative tra i presidenti degli enti e i funzionari ministeriali, che gestiscono le procedure di finanziamento chiamate ipocritamente «premiali», ma di fatto discrezionali. Le decisioni si spostano dai laboratori ai palazzi. Le cifre parlano chiaro. Il finanziamento in corso dei bandi di ricerca per tutti gli atenei e per l'insieme delle discipline accademiche è ridotto a 30 milioni di euro all'anno. Ma non si dica più che il debito non consente di fare meglio, perché i soldi ci sono quando si tratta di evitare i bandi: sei volte tanto (oltre 180 milioni di euro) sono assegnati a un solo ente, appunto la Fondazione IIT, che poi distribuisce finanziamenti agli atenei e ottiene, in cambio, la firma delle pubblicazioni scientifiche, migliorando immeritatamente il suo *ranking*. Per consolidare questo sistema i Governi hanno sempre impedito, negli ultimi anni, la costituzione di una moderna Agenzia della ricerca, nonostante le proposte venute dalla comunità scientifica e gli indirizzi approvati dal Parlamento. Ricordo, a tale proposito, la risoluzione della Commissione 7a. L'Agenzia consentirebbe un libero confronto di idee e di progetti, entro una ben definita politica nazionale ed europea; avrebbe il compito di diffondere i bandi per i progetti, di eliminare i conflitti di interesse

Che cosa impedisce, allora, l'istituzione dell'Agenzia della ricerca? È sotto gli occhi di tutti che l'ostacolo è la resistenza del Ministero

È sotto gli occhi di tutti: problemi come la manutenzione delle scuole, che dovrebbero essere risolti in via ordinaria, con la buona amministrazione, vengono portati in Parlamento per ottenere il sigillo della legge a provvedimenti emergenziali;

addirittura per decreto-legge, di una nuova università, senza ricorrere a provvedimenti ordinari e di programmazione. È necessaria - come dimostra anche questo decreto-legge - una profonda riorganizzazione del Ministero, affinché la struttura si concentri sulla politica dell'istruzione e rinunci alle competenze nella politica della ricerca, che invece possono essere utilmente affidate a una moderna Agenzia, guidata da prestigiosi scienziati, scegliendo il modello delle migliori esperienze internazionali*.

più urgente per il Paese, ovvero le modifiche al codice penale per l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e le disposizioni in materia di trasparenza quella sì necessaria - e contrasto alla corruzione. Avete votato contro senza neanche voler utilizzare il sistema elettronico. questo provvedimento che voi ritenete urgente, al primo punto autorizza la spesa di ulteriori 64 milioni di euro per assicurare fino al 30 novembre 2016 gli interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, continuando a utilizzare quelle imprese che già forniscono servizi di pulizia nelle scuole e chiedendo alle stesse di rispettare condizioni economiche e tipologie di strumentazioni relative all'appalto

una scelta, la vostra, in linea con la logica emergenziale e senza carattere risolutivo, che lascia in uno stato di ulteriore incertezza l'intero settore dei servizi di pulizia e ausiliari destinati alle scuole. Già nell'ottobre 2014 un'inchiesta su «il Fatto Quotidiano» svelò l'impronta prettamente clientelare e di facciata del programma scuole belle voluto e venduto al Paese dal Governo Renzi come interventi di manutenzione degli edifici scolastici: colleghi, 150 milioni di euro per il 2014, 450 milioni fino ai primi mesi di quest'anno sono stati distribuiti tra le varie province del Paese non sulla base degli interventi richiesti con urgenza dagli istituti o, in alcuni casi, neppure voluti. I dirigenti sono stati costretti ad accettare questi fondi,

La precarizzazione del personale ATA e degli ex lavoratori socialmente utili è, infatti, diretta conseguenza delle politiche annose di esternalizzazione adottate negli ultimi anni per i servizi di pulizia nelle scuole. Con il sensazionalistico programma scuole belle di Renzi si è giunti, con pochissime ore di aggiornamento, addirittura all'aberrazione dell'impiego, sempre più consistente e vergognoso, di donne di mezza età,

un ruolo importantissimo per il funzionamento delle scuole pubbliche. Oltre al peggioramento della condizione e dei salari dei lavoratori, le esternalizzazioni non hanno prodotto alcun risparmio, continuando a favorire le cooperative

Era urgente fare ciò che noi abbiamo più volte detto, sia alla Camera che al Senato e anche in Commissione, invitandovi ad affrontare seriamente sicurezza e pulizia nelle scuole, perché è un problema - quello sì - da affrontare con urgenza.

di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. Istituito con legge n. 35 del 2012, il Gran Sasso Science Institute potrebbe rappresentare per il territorio abruzzese, almeno sulla carta, un importante volano di sviluppo, capace di portare positive ricadute sul territorio grazie all'ambiziosa *mission* che si prefigge, cioè attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione fra ricerca e impresa. Tale progetto, però, è stato finora capace solo di attrarre cospicui fondi: 36 milioni di euro per il triennio 2013-2015, più ulteriori 9 milioni di euro, già assegnati con l'ultimo decreto milleproroghe, ai quali si vanno ad aggiungere i 18 milioni di euro assegnati con la delibera CIPE 76/2015 per il triennio 2016-2018. Premesso che non c'è chiarezza sull'utilizzo di questi fondi, non si può non fare una riflessione più ampia sulla condizione in cui versa la ricerca scientifica nel nostro Paese, dove alla dispersione, all'inaffidabilità, all'intermittenza e alla scarsa trasparenza con cui vengono assegnate le risorse, alla quasi totale assenza di verifiche *in itinere* o *ex post* dei risultati raggiunti, alle sistematiche sforbiciate ai fondi destinati alla ricerca fanno inspiegabilmente da contraltare progetti ambiziosi e dispendiosi, come appunto il Gran Sasso Science Institute o o il "petaloso" Human Technopole, che dovrebbe sorgere addirittura nell'ex area dell'Expo; e dovremmo prima capire i fallimenti che ci sono stati in quell'area

e costanza con le quali vengono invece stanziate tali risorse, alla luce dei tagli registrati nel comparto della ricerca universitaria negli ultimi anni. Questo ancora non ci è dato di capire. Ritengo che una tale schizofrenia attesti la tendenza della politica negli ultimi anni a considerare la ricerca scientifica e la scuola non come le vere priorità per lo sviluppo del nostro Paese, bensì come il terreno sul quale far crescere, attraverso continui *spot*,

Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, il decreto-legge che andiamo a convertire va a rafforzare positivamente il progetto della buona scuola e definisce meglio un'idea di Paese che punta sul merito, sulla cultura, sulla ricerca e sull'educazione di tutti, ma soprattutto dei giovani cittadini. Nella buona scuola, checché ne dica qualcuno, ci sono moltissime cose positive, che si stanno puntualmente realizzando. Sconfitti sono stati il disfattismo degli apocalittici e e il qualunquismo di molti colleghi, che avevano presunto un quadro drammatico: nulla di tutto questo. La buona scuola funziona e funziona bene. Può e deve essere migliorata, e siamo qui anche per questo. Le assunzioni stanno andando avanti, l'alternanza scuola-lavoro sta funzionando, l'autonomia scolastica è rafforzata e tanto altro. Con questo decreto-legge si vanno ulteriormente a rafforzare alcune misure e bene ha fatto la relatrice Francesca Puglisi, che ringrazio, a sottolinearne l'importanza. Fondamentali sono la prosecuzione e il rifinanziamento del programma scuole belle ed è assolutamente inaccettabile che esso venga svilito. di un programma importante, che questo Governo ha realizzato per la prima volta, dopo anni di indifferenza. Posso dirlo, perché sono stata assessore comunale alla scuola e Presidente di Provincia e ho avanzato numerose

L'inclusione sociale si persegue con i fatti e non con le chiacchiere e l'emendamento del Governo che ha allargato il *bonus* ai diciottenni con permesso di soggiorno è una misura giusta e civile, che non crea discriminazioni. La *card* di 500 euro è parte della risposta italiana al terrorismo e alla mafia: incentivare i giovani alla cultura è un modo per educare alla tolleranza, alla responsabilità e alla legalità. Si tratta di un principio che vale per i diciottenni italiani, ma anche per gli altri che vivono nel nostro Paese. Antonino diceva che la mafia non ha paura della giustizia, ma ha paura della scuola e noi dobbiamo fare in modo che la scuola sia sempre di più un deterrente all'illegalità, alla mafia e al terrorismo. Diversamente dalla collega che ha parlato poco

Ringrazio tutti, perché solo poche settimana fa, durante la visita importante del Presidente del Consiglio ai laboratori di fisica nucleare fu assunto un impegno, che è stato

Si tratta di uno dei progetti di rafforzamento dell'alta formazione e della ricerca scientifica italiana, tra i più innovativi e avanzati realizzati negli ultimi decenni. Illazioni su questa struttura fanno solo male alla città che la ospita, ovvero L'Aquila,

questa struttura è stata resa possibile proprio grazie all'impulso dell'OCSE, che ce l'ha indicata come uno dei progetti strategici per il rilancio della città terremotata e di tutto il cratere, che non può solo essere ricostruita, ma deve guardare lontano, investendo sulla ricerca e sull'innovazione.

facoltà scientifiche. Operando in sinergia con tali istituzioni e attivando collaborazioni con istituti di ricerca e alta formazione nazionale e internazionali, il GSSI sta favorendo l'attrazione di risorse di eccellenza nel campo della ricerca e della imprenditorialità innovativa. Quattro i corsi di dottorato attivati: fisica, matematica, informatica e sviluppo territoriale. Altro che chiacchiere! Nel primo triennio, oltre tremila sono state complessivamente le domande ricevute da tutto il mondo, per un totale di circa 150 allievi di dottorato e giovani ricercatori selezionati, di cui circa il 50 per cento provenienti dall'estero. Non mettiamo in fuga i cervelli, ma, anzi, attraiamo cervelli da altri Paesi. Una realtà nata dopo il terremoto secondo un piano strategico preciso. Di nuovo ringrazio ed esprimo grande soddisfazione per la stabilizzazione e il riconoscimento nel sistema universitario della Scuola sperimentale di dottorato internazionale GSSI, per il riconoscimento delle sue attività e per il giusto, adeguato finanziamento alle attività. Così si aiuta la ricerca in Italia e si rende il Paese più competitivo e si aiuta a crescere e a valorizzare un territorio che non vuole più pensare alle macerie, ma vuole guardare, anche con questi progetti, a un futuro importante, fatto di competitività, di impegno sugli studenti, di studio e di e di ricerca. Le previsioni non sono state smentite e per questo, con orgoglio, voterò a favore di

e della ricerca, che con l'articolo 2 stabilizza e riconosce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. Questo disegno di legge tratta della programmazione e della funzionalità della ricerca e in questa discussione generale vorrei perciò soffermarmi sull'improvvisazione della vicenda dello Human Tecnopole, su cui ho presentato un apposito ordine del giorno, il G2.1. Vicenda che è stata oggetto anche delle riflessioni di alcuni senatori, in 7a Commissione e anche in Aula stamattina, e tra loro voglio ricordare i senatori Tocci e Bocchino. vicenda è esemplare delle criticità delle procedure che governano la ricerca in Italia e della possibilità - se lo volessimo e ci impegnassimo a farlo - di muovere passi da gigante proprio per migliorare la funzionalità del delicato ecosistema della ricerca pubblica di cui si parla nel disegno di legge. Per parlare del Tecnopolo, vorrei prima partire dal vincolo etico che lega ogni studioso di ogni disciplina ai cittadini che con le loro tasse sostengono quegli studi, vincolo che implica per lo studioso l'impegno a essere onesto, cioè a riportare e rispettare le prove, ad essere trasparente e a mettere in atto ogni comportamento affinché ogni idea razionale possa essere liberamente messa a confronto con ogni altra, nel pieno diritto ad essere valutata. È attraverso questo meccanismo, che implica libertà e uguaglianza delle idee per l'accesso alle risorse pubbliche su base competitiva, che si restituirà al cittadino la miglior proposta sostenibile con i fondi pubblici. Di scorciatoie non ne esistono. È un metodo questo che nulla ha a che fare con le necessità e con le contingenze o convenienze politiche, ma che orienta ogni decisione e valutazione sulla selezione delle idee migliori e sul controllo dei fatti. Adottare queste regole significa rispettare la struttura etica della scienza e rispettare l'impegno verso i cittadini. Questo è quel che si chiede alle comunità scientifiche nei Paesi liberi, democratici ed economicamente avanzati. La stessa richiesta rivolgo a noi, come decisori politici, e al Governo. La mia richiesta è che si tuteli lo spazio di libertà delle idee di tutti, dei giovani e dei meno giovani, piccole o grandi che siano, messe in competizione tra loro, perché le idee più belle possano tradursi in un miglior futuro per tutti. Nel nostro Paese abbiamo molti problemi irrisolti sul fronte ricerca. Il finanziamento pubblico alla ricerca e ancora di più alla ricerca di base, che studia in piena dignità per capire e consegnare conoscenza a tutti noi, è irrisorio, discontinuo, frammentato, spesso inaffidabile. Succede anche che gli stessi obiettivi di ricerca siano distribuiti su più erogatori pubblici. Succede che ai bandi Prin del MIUR non possono accedere direttamente gli studiosi del CNR e che ai bandi del Ministero della salute non possono applicare gli studiosi universitari: i bandi del CNR sono per il solo CNR e così via e spesso gli obiettivi sono gli stessi. Dovremmo rimuovere questa frammentazione, unificare gli obiettivi e avere, al contempo, una garanzia di valutazione di ciò che viene finanziato con soldi pubblici. Ammetto che non riesco più ad ascoltare giovani e meno giovani dirmi che se non si è parte del potentato amicale giusto - intendo di scienziati e studiosi si avrà il finanziamento pubblico; che se si denunciano le anomalie si verrà esclusi per gli anni a venire; che se si tace, si avrà una piccola parte, garantendola più cospicua ad altri. È anche da queste modalità corruttive del metodo della scienza, oltre che dell'etica pubblica, che gli studiosi scappano. C'è un modo per superare queste distorsioni. Basterebbe guardare ai Paesi che ci stanno accanto e dar vita a un'Agenzia nazionale per la ricerca, mutuando i modelli già esistenti in Spagna, Francia, e, con sistemi più complessi ed efficaci, in Germania e Gran Bretagna, adattandoli alle peculiarità dell'Italia. Gentili colleghi, la ricerca pubblica in tutte le discipline del sapere ha bisogno di cinque componenti: continuità dei bandi presso i quali competere, perché un'idea che cresce non funziona ad intermittenza; procedure affidabili e granitiche, unificate nel metodo e diversificate in funzione degli obiettivi; valutazioni terze, indipendenti, competenti; controlli ferrei ad ogni passaggio; rendiconti certi e verificabili su cosa viene finanziato e su cosa si è generato. L'Agenzia nazionale per la ricerca deve essere questo. Progettare un simile ente potrebbe non comportare grosse spese per lo Stato. Si potrebbe pensare a reindirizzare finanze e risorse umane frammentate tra i vari enti governativi, per concentrare in un'unica struttura funzioni duplicate in diversi uffici. Inoltre, si potrebbero ridurre o sospendere per qualche anno i flussi dei finanziamenti pubblici a enti poco efficienti oppure a quelli che hanno già accumulato un tesoretto di denaro pubblico, ora accantonato. nazionale per la ricerca nascerebbe come distinta dalla politica, cui spetta la decisione degli obiettivi da perseguire e delle risorse da assegnare ma che non può scegliere discrezionalmente chi finanziare. Necessariamente, l'Agenzia per la ricerca deve essere ben distinta dalla comunità degli studiosi che poi eseguiranno le ricerche. Penso all'Agenzia come ad una casa di cristallo e come ad un passo in avanti per vederci ancora più chiaro circa le norme sulla gestione dei fondi pubblici in Italia in un settore dove i risultati sono ben monitorabili. Le sue funzioni devono includere l'allestimento di ogni sensibile procedura per garantire al cittadino che i suoi soldi siano ben spesi, ripristinando fiducia nelle istituzioni. La costruzione di una simile agenzia nel nostro Paese si rende anche più urgente oggi, in vista della realizzazione del progetto Human Technopole*,* il polo tecnologico dedicato alle scienze della vita e alla nutrizione che il Governo ha annunciato di voler creare nell'area dell'Expo, impegnandosi a garantire 1,5 miliardi di euro in dieci anni. Un progetto nato in modo improvvisato come non avviene in nessun Paese, che l'Esecutivo ha affidato a un ente, l'Istituto italiano di tecnologia, scelto arbitrariamente come perno dell'operazione senza competizione pubblica, quindi operando scelte discrezionali contro ogni logica di massimizzazione dell'investimento pubblico e contro il metodo della scienza. Si tratta di un ente al quale, senza alcun bando pubblico, sono già stati destinati per legge 80 milioni di euro senza controllo e senza un fine chiaro. Ecco che, nel tentativo di dare risposte agli interrogativi emersi dopo l'annuncio del Governo, ho condotto un'analisi, basandomi su dati pubblici e i cui primi risultati sono stati raccolti in un documento di studio di circa 50 pagine per il Parlamento e i cittadini che la scorsa settimana ho depositato qui in Assemblea, anche in vista dei prossimi passaggi parlamentari. Lascio a voi l'eventuale approfondimento di quel documento, ma vorrei qui riassumere quattro conclusioni a cui sono giunta e che dimostrano come la dinamica della vicenda Human Technopole sia paradigmatica di come la ricerca pubblica non debba essere promossa. La prima conclusione si basa sulle esperienze storiche e sulle analisi politico-economiche, che dimostrano che è un errore stabilire per legge quale idea e progetto scientifico sostenere. Sul Tecnopolo milanese sono sbagliate le premesse, perché nella scienza, come nel settore degli appalti pubblici, ogni assegnazione di fondi pubblici non può prescindere da una competizione per sostenere le migliori proposte e i migliori enti proponenti. Come seconda conclusione, nel documento si evidenzia come le stesse esperienze e analisi dimostrino che la concentrazione continuativa e non competitiva di denaro pubblico per la ricerca in poche mani sia inefficace. luogo, chi riceve denaro pubblico deve rendicontare pubblicamente. L'assegnazione continuativa di ingenti somme di denaro pubblico a modelli organizzativi di centri di ricerca come l'Istituto Italiano di Tecnologia fondazione di diritto privato largamente finanziata con fondi statali, che si sottraggono alle rendicontazioni pubbliche e all'amministrazione trasparente, non rispetta l'obbligo etico di fornire prove adeguate della ricaduta dell'investimento e, a mio avviso, non è il modello di *governance* da implementare nel Tecnopolo milanese. Infine, l'ente beneficiario scelto come coordinatore del Tecnopolo non ha le competenze specifiche negli ambiti indicati dal Governo come contenuti per il centro di ricerca, scienze della vita e nutrizione. Ciò ha portato l'ente a reclutare altrettanto arbitrariamente, quindi in modo discriminatorio, tematiche, enti e studiosi. È su queste basi che ho presentato l'ordine del giorno che - mi rendo conto - in caso di apposizione della fiducia non potrà essere discusso, auspico comunque il Governo voglia esprimersi. Vorrei invitare l'Esecutivo a ripensare le strategie per la realizzazione del progetto Human Technopole e, soprattutto, ad adottare ogni atto necessario e opportuno realizzare un percorso trasparente e scientificamente e culturalmente partecipato e competitivo sull'esempio di esperienze all'estero, valide e di successo. Esistono esempi, su cui mi soffermo nel documento Credo che ripensare la strategia su Human Technopole e farlo a valle della realizzazione di un'Agenzia nazionale per la ricerca sarebbe davvero un cambio di passo e un segno dell'impegno del Governo a voler lavorare nell'ottica di una più completa e funzionale riforma del sistema di finanziamento della ricerca in Italia.

che sono risultati vincitori di un'esercitazione di *drafting* legislativo svolta sotto la supervisione degli Uffici del Senato, nell'ambito dell'insegnamento «La lingua del diritto».

Signor Presidente, in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto - in modo particolare, nell'intervento di particolare impegno e autorevolezza della senatrice Cattaneo - sono state sollevate questioni di grande importanza relative alla politica della ricerca scientifica. Si tratta di questioni di interesse vitale per il mondo stesso

Naturalmente mi rendo ben conto che il provvedimento di cui stiamo discutendo tocca solo tangenzialmente questa materia, attraverso l'articolo citato anche dalla senatrice Cattaneo, e su cui si è soffermato

Ma la verità, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, è che non ci sono state altre sedi per informazioni e chiarimenti che avrebbero dovuto essere offerti al Parlamento. oggi, in modo particolare, si tocca il problema del progetto Human Technopole, destinato a realizzarsi nell'area ex Expo. Si tratta di un progetto cui bisogna guardare positivamente, sapendo che può rappresentare qualcosa di serio e significativo per lo sviluppo ulteriore della ricerca, in modo particolare in quei campi che sono stati designati quasi come tema dell'Esposizione universale realizzatasi a Milano. Noi abbiamo avuto una decisione di Governo e un annuncio nello scorso novembre attraverso la presentazione di un decreto-legge, poi convertito in legge con votazione, credo, della fiducia in Parlamento o, almeno, al Senato; decreto con cui sono stati stanziati 80 milioni per la presentazione di un progetto per la struttura Human Technopole da realizzare in quella area da parte dell'Istituto italiano di tecnologia, sentite le tre università milanesi. è avvenuto lo scorso novembre. Poi è accaduto che, aprendosi la discussione fuori dal Parlamento (in Parlamento non se ne è mai potuto discutere), sono stati fatti molti rilievi polemici cui ha risposto lo stesso Istituto italiano di tecnologia con un suo comunicato ufficiale il 27 marzo scorso. si dava notizia di aver già presentato ai Ministri competenti la proposta di progetto in data 25 febbraio. Oggi siamo a metà maggio o quasi e i seguiti di quella di quella decisione-annuncio non sono mai stati chiariti. Non c'è stata alcuna informazione. In quello stesso comunicato che ho appena citato si dice che sarà consultato o che è in via di consultazione (e una consultazione c'è già stata ed è terminata, ma non se ne sa nulla) un *panel* internazionale, la cui composizione non è mai stata resa nota. Né tanto meno è stato reso noto

da esperienze internazionali note a quanti si occupano dei problemi della ricerca scientifica. Io credo che bisogna dare soddisfazione ai problemi posti dalla senatrice Cattaneo nel suo ordine del giorno, nonostante l'apposizione della questione di fiducia sulla conversione di questo decreto.

che nella sua replica si dicano cose precise, si assumano degli impegni chiari, sia nel senso di fornire tutte le informazioni che sono mancate, sia di mostrare una disponibilità, che io non posso immaginare non vi sia da parte del Governo, a ripensare decisioni frettolose che sono largamente discutibili sul piano del metodo e su quello degli interessi generali della ricerca scientifica e dunque del futuro del nostro Paese.

Qualcuno ha parlato di un altro tassello importante della riforma della scuola; qualcun altro ha enfatizzato la portata di questo decreto che, al di là dell'articolo riguardante dell'articolo riguardante il centro del Gran Sasso, si occupa essenzialmente di piccole cose.

In materia di funzionalità del sistema scolastico troviamo appunto le disposizioni dell'articolo 1, che sono destinate essenzialmente alla proroga dei servizi scolastici di pulizia e ausiliari

disposizione in un linguaggio più pragmatico e chiaro, si tratta di quello stillicidio che riguarda quella platea di lavoratori socialmente utili che da anni

delle responsabilità, nonché più complicate dal punto di vista della formazione di questo personale, vengono risolte con altri tipi di attività, per lo più demandate agli enti proprietari di queste scuole

oltre al garantire il prosieguo delle attività lavorative di questo personale, semplicemente per fare piccoli interventi di tinteggiatura o piccolissime e banali manutenzioni. Non ci si pone il problema, quando si parla di funzionalità del sistema scolastico, che le scuole hanno ogni giorno altre esigenze, ben più urgenti. Si è fatto tanto, nel corso degli ultimi anni, utilizzando anche in modo cospicuo fondi europei per informatizzare le scuole. le scuole. La maggior parte delle scuole iniziano ad avere lavagne interattive multimediali che, dopo qualche mese di funzionamento, proprio perché sono strumentazioni di certa complessità, spesso non funzionano più ed i dirigenti scolastici non hanno i fondi per poterle riparare. Queste lavagne comportano, ad esempio, che le scuole debbano essere dotate di un collegamento Internet veloce e sempre funzionante, mentre la rete *wi-fi* nelle scuole spesso non funziona o funziona male e gli interventi per il ripristino sono delle delle vere e proprie acrobazie, che i dirigenti scolastici cercano di fare o con fondi inesistenti o rimettendosi alla buona volontà e alla collaborazione dei sindaci, che purtroppo non sempre hanno nei loro bilanci

di provvedimenti tampone, che si sovrappongono di mese e mese e di anno in anno. Cosa dire, peraltro, a proposito di funzionalità del sistema scolastico e di buona scuola, dei primi fondi che i dirigenti scolastici stanno prime settimane per la valutazione del merito dei docenti? Criteri difficilissimi da introdurre, lunghissime e serotine discussioni

dei docenti, oppure ad ingessare la situazione in uno *stand by*, per cui il dirigente scolastico, con la commissione che magari si nomina all'uopo, non riesce a trovare dei criteri pienamente convincenti.

solo al personale docente o agli insegnanti di sostegno. Questa è una battaglia di civiltà che, quando si adottano decreti d'urgenza, bisognerebbe porsi e non rimandare di volta in volta. Registro, se dovesse andare in porto, che l'emendamento sulla scuola dell'infanzia è l'unica nota positiva di questa pagina tormentata del decreto-legge

Il 17 febbraio ho presentato, insieme ad altri colleghi, un'interrogazione in cui ponevamo il problema che le Province sono titolari al momento, con la legge vigente, la n. 56 del 2014, della gestione della sola edilizia scolastica. di questo presupposto ho evidenziato che non è stata quindi riproposta la vecchia e più ampia funzione amministrativa, attribuita dall'articolo 14, comma 1, lettera *i),* della legge n. 142 del 1990 e mantenuta dall'articolo 19, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo n. 267 del 2000, il testo unico degli enti locali. Con quella interrogazione chiedevamo al Governo di chiarire che, oltre alla gestione dell'edilizia scolastica, bisognava porsi il problema di tutte le utenze, di tutte le spese ordinarie che non competono più alle Province e che dovrebbero competere ai dirigenti scolastici, quindi al

se ben ricordo, quando il Presidente del Consiglio venne in Aula la prima volta ci disse che la scuola per lui - e quindi penso anche per questa maggioranza - doveva essere la priorità.

da quando abbiamo iniziato a trattare il provvedimento in esame, il Ministro non si è mai visto. Guardate i banchi del Governo: del Ministro neanche l'ombra. È talmente una priorità che nemmeno il Ministro viene in Aula a parlare delle priorità di questo Governo! Montevecchi)*. È talmente una priorità che questa maggioranza e questo Governo - ormai la voce gira ed è sempre più insistente - hanno deciso di tarpare le ali ancora una volta al dibattito parlamentare, dal momento che si intende mettere la fiducia.

da trattare: 40 emendamenti. Mettete la fiducia su un provvedimento che teoricamente sarebbe andato via tranquillo,

Significa che questo provvedimento è una rottura di scatole, che per questa maggioranza e per questo Governo deve essere fatta fuori il più velocemente possibile: diciamoci le cose come stanno! Oppure nel provvedimento in esame avete inserito talmente tante stupidate che forse è meglio mettere la fiducia per farlo approvare il più velocemente possibile, per non rischiare eventuali situazioni imbarazzanti in Aula. Signor Presidente, l'estate scorsa avevamo la buona scuola, adesso abbiamo le scuole belle. Sul

Questo provvedimento, signor Presidente, è un altro strumento per far vedere al popolo, distratto in altro, che il signore di Firenze sta facendo qualcosa: dimostriamo che sulla scuola Renzi sta facendo qualcosa. Nel frattempo, colleghi, le scuole sono obsolete ed è sotto gli occhi di tutti che cadono a pezzi:

risparmiare anche sul riscaldamento. Ma per Renzi le scuole sono belle, sono bellissime, colleghi. In cosa consiste, quindi, il programma scuole belle? Consiste in interventi di facciata per dare sempre più soldi a quelle cooperative amiche degli amici degli amici degli amici.

perché oltre non si può toccare. Ma non si può neanche scrostare la tinteggiatura che c'era prima, quindi si dà pittura su pittura: diamo una mano di vernice, così almeno facciamo vedere che qualcosa facciamo, tanto i cittadini italiani sono distratti da altro e Renzi fa vedere che le scuole sono belle.

e non un interessamento reale ai lavoratori, come riportato nel testo («al fine di assicurare la continuità occupazionale e reddituale» dei lavoratori impegnati). Reddituale? Per non essere prolisso, do alcune indicazioni.

cari colleghi, costa molto di più che assumere direttamente collaboratori scolastici (i bidelli), i quali, oltre a fare le pulizie, si occupano anche di accoglienza, sorveglianza, assistenza, cosa che i dipendenti di Manutencoop, che noi paghiamo profumatamente, non possono fare per contratto. Terzo, ma non ultimo punto: i lavoratori assunti non percepirebbero uno stipendio dignitoso, considerato che attualmente, con il loro lavoro, devono guadagnare soprattutto i caporali legalizzati, i quali individuano unicamente le persone da mandare nelle scuole, mentre la loro organizzazione spetta alle scuole stesse. di un caporalato gestito dallo Stato italiano. Faccio un esempio di quanto paga una scuola un bidello a Manutencoop: 4.800 euro, per un mese. Pensate che al dipendente arrivino 4.800 euro per un mese di lavoro? Al dipendente arrivano meno di 1.000 euro. Questo è quello che paga lo Stato italiano per avere un servizio scadente da chi ci sta offrendo servizi scadenti, cari colleghi. Oltre a questa problematica,

umiliato gli insegnanti che operano da anni nel mondo della scuola e che oggi si vedono scavalcati da chi la scuola nemmeno la conosce; oppure costretti a dimostrare, con un concorso farsa (che fa acqua da tutte le parti e lo stanno dicendo tutti), di essere in grado di insegnare. Persone che insegnano da anni sono costrette a dover fare un concorso e vengono parificate ad altre che la scuola non l'hanno mai vista. Questa è la buona scuola di Renzi.

perché questa persona, purtroppo, ha la "sindrome dell'annuncite" e deve raccontare sempre al mondo le cose che vuole fare e che poi non è in grado di fare. Cari colleghi

È una lettera dai contenuti preoccupanti ed allarmati dove si ratifica una insufficienza grave dell'organico a disposizione degli uffici a cui si è oggettivamente impossibilitati a rimediare con palliativi sostitutivi così come si è proceduto a fare sino ad oggi e da troppo tempo. Questo dato, assolutamente preoccupante, riguarda nello specifico la procura di un territorio mai come oggi particolarmente delicato e sensibile. Bari, infatti, sta vivendo una vera e propria recrudescenza dell'azione di gruppi criminali. Bari è il luogo dove un paio di giorni fa è stato rinvenuto oltre mezzo chilo di tritolo destinato probabilmente ad un attentato al procuratore di Napoli. Bari appare sempre più come una possibile zona di copertura e di snodo per il transito e lo stazionamento di terroristi e sospettati tali. Un insieme di dati, quindi, che lascia ancor più preoccupati per il fatto che si associano ad un più vasto e diffuso stato di agitazione e mobilitazione che gli operatori della giustizia di questa Regione, della mia Regione, la Puglia, vivono da tempo, in ragione della paventata riforma della geografia giudiziaria. Una riforma che vorrebbe la chiusura di alcuni presidi fondanti dello Stato, ad esempio la corte d'appello di Lecce, e con essa la relativa dismissione della direzione distrettuale antimafia, nel pieno dunque di un processo di mafia - sì, proprio di mafia - contro una possibile nuova germinazione della SCU. Faccio riferimento al processo Eclissi, dove gli indagati hanno ricusato gli avvocati, affermando testualmente che la SCU non esiste e nessuno deve più dubitare. Ma altri dubbi insistono, anche sulla stessa concentrazione e dislocazione degli uffici del tribunale di Bari, ritenuti ormai al collasso e del tutto incapaci di far fronte alle reali esigenze cui questa istituzione deve far fronte. Chiedo pertanto a lei,

che ha sede nel Comune di Molteno e che produce catene da neve. Lo scorso anno è stata acquisita da una multinazionale austriaca, la Pewag; alla vigilia del 1º maggio, questa società ha deciso di chiudere lo stabilimento lecchese e di delocalizzare la propria produzione in Carinzia e nella Repubblica ceca. dipendenti sono a forte rischio di licenziamento; i motivi sono le alte tasse e l'alto costo dell'energia (quindi l'alto costo del lavoro) e l'alta burocrazia.

così come ho fatto la scorsa settimana con l'interrogazione 4-05745, perché sono successe due novità. La prima è che abbiamo scoperto che, con il famoso *jobs act* che il *premier* Renzi continua a decantare, nel caso delle società che delocalizzano e chiudono non ci sono più gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, ovverosia questi centotrenta dipendenti lecchesi finiranno direttamente in mobilità, senza beneficiare

il ministro Calenda, al quale mi ero già rivolto la scorsa settimana e che invito caldamente a convocare un tavolo istituzionale con la proprietà e con i rappresentanti sindacali, perché il problema della König, che è un problema generale, venga affrontato. Deve essere assolutamente scongiurata la chiusura di questa società, invitando eventualmente la proprietà a presentare un piano industriale per una riconversione della produzione. Lo scandalo è che il *jobs act* lascia per strada i dipendenti della König, così come lascerà per strada i dipendenti di altre società acquistate in questi mesi da società estere per rubare il marchio e per lasciare solo terra bruciata nel nostro territorio italiano. *(Applausi del